Sarà proclamato eletto colui che otterrà la maggioranza assoluta dei voti dei componenti del Senato. Per le operazioni di voto è stata predisposta un'urna che, una volta esaurita la chiama, resterà ordine alfabetico, potranno passare sotto il banco della Presidenza, comunicando ai senatori Segretari il proprio nome, e deporre la scheda nell'urna predisposta. Dichiaro pertanto aperte le operazioni di voto a scrutinio segreto e invito i senatori Segretari a procedere alla chiama.

Boccardi, Bocchino,

Dalla Tor, Dalla Zuanna,

De Petris, De Pietro,

De Pin, De Poli,

Guerrieri Paleotti Ichino,

il decreto-legge n. 50 del 2017 riveste una particolare importanza nell'attuale fase congiunturale, in quanto oltre ad assicurare il controllo dei conti pubblici, promuove, attraverso un articolato insieme di misure, interventi per accompagnare la crescita dell'economia e dell'occupazione nel nostro Paese. Il sentiero su cui si sviluppa il provvedimento è stretto. La priorità degli interventi è quella di ridurre l'indebitamento come concordato con l'Unione europea. Tuttavia, a fronte dello sforzo richiesto al nostro sistema economico, sono state predisposte e rafforzate, durante il dibattito parlamentare, numerose disposizioni volte alla disattivazione delle clausole di salvaguardia e alla riduzione dell'impatto della manovra su imprese e cittadini. A questi interventi sono state affiancate altre importanti ed attese disposizioni tra le quali si segnalano misure per gli enti territoriali e per il terremoto. La prima parte del decreto-legge in esame contiene le misure volte al controllo dei conti pubblici. L'intervento correttivo è complessivamente pari, in termini di indebitamento netto, a circa 3,1 miliardi di euro ed è in gran parte operato sul lato delle entrate, per circa 2,8 miliardi di euro, ed in parte residuale, per poco meno di 0,3 miliardi, sul lato della spesa.

In tale contesto, particolare rilievo assumono le misure volte al contrasto dell'evasione fiscale, quali l'estensione dello *split payment* alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle amministrazioni le modifiche all'esercizio del diritto alla detrazione IVA, il contrasto alle compensazioni indebite, la rideterminazione delle aliquote dell'aiuto alla crescita economica (ACE), le nuove disposizioni sul pignoramento. Si tratta di misure che per un verso aumentano la pressione sul sistema produttivo in rapporto all'introduzione di nuove disposizioni sullo *split payment*, ma che peraltro sono state adottate con adeguate contropartite. Ad esempio, sul tema liquidità delle imprese è stata adottata una misura che riduce in modo molto significativo i tempi per il rimborso dei crediti vantati nei confronti della pubblica amministrazione in termini di compensazione. A queste si aggiungono le misure volte a deflazionare il contenzioso tributario, tramite l'innalzamento della soglia della mediazione nelle controversie tributarie e l'introduzione di modalità agevolate per le liti pendenti. Alle proposte originarie del decreto-legge relative alla parte fiscale sono state aggiunte durante l'esame alla Camera ulteriori misure come l'introduzione della cosiddetta *web tax*, che va ad interessare società non residenti in Italia che appartengono a gruppi multinazionali che effettuano cessioni di beni e servizi in Italia per un ammontare superiore a 50 milioni di euro annui, le quali potranno avvalersi di una procedura di cooperazione e collaborazione con l'Agenzia delle

che incrementano e rimodulano la tassazione sui tabacchi e le disposizioni sui giochi, con le quali si dà attuazione in maniera organica al piano di riduzione del numero degli apparecchi per il gioco. Sempre dal lato delle entrate, è importante richiamare l'introduzione di indici sintetici di affidabilità fiscale dei contribuenti, a cui sono correlati benefici specifici in relazione ai diversi livelli di affidabilità del contribuente, migliorando la collaborazione tra questo e l'amministrazione finanziaria.

Per effetto degli interventi sul lato delle entrate, il provvedimento prevede la parziale disattivazione delle clausole di salvaguardia, prefigurando un percorso che riduce, da oltre 19 miliardi a poco più di 15 miliardi di euro, la correzione di base che dovrà essere adottata in sede di legge di bilancio per l'anno 2018 per sterilizzare il previsto aumento - da evitare - dell'IVA e delle accise. A fronte delle misure di correzione dei conti pubblici, il provvedimento prevede una serie di misure finalizzate al rilancio economico e sociale del Paese. Tali interventi si sviluppano su quattro aree prioritarie di intervento: i trasporti, il lavoro, il sostegno alle imprese e ai contribuenti e gli investimenti. Particolare rilevanza assumono le disposizioni sul trasporto ferroviario, tra le quali si segnalano gli interventi relativi alla gestione delle reti ferroviarie regionali, le disposizioni per il completamento del Programma grandi stazioni; l'autorizzazione delle attività propedeutiche all'avvio dei lavori della nuova linea ferroviaria Torino-Lione; lo sviluppo, da parte di ANAS SpA, di opportune sinergie con il gruppo Ferrovie dello Stato e per il trasferimento a Ferrovie dello Stato Con specifico riguardo al trasporto aereo, si segnala l'introduzione nel provvedimento delle disposizioni finalizzate a garantire la continuità operativa dell'Alitalia già contenute nell'apposito decreto-legge all'esame della Camera. particolare rilevanza assumono le disposizioni nate nel dibattito parlamentare che introducono una nuova disciplina delle prestazioni di lavoro occasionale che va a colmare il vuoto lasciato dall'abrogazione della disciplina Nessuno può negare l'utilità e la necessità che tra i contratti di lavoro disponibili in Italia ci sia anche un contratto che regoli il lavoro occasionale. Il contratto, diversamente dal passato, deve contenere certezza di doveri e di diritti per entrambe le parti, in piena trasparenza e totale tracciabilità. In sintesi, viene introdotta una nuova forma di contratto di lavoro, che ha caratteristiche trasparenti e che rende il datore e il lavoratore rispettivamente titolari di doveri e di diritti. forma di contratto di lavoro va a colmare un'esigenza espressa dalle famiglie, dalle imprese e dagli stessi lavoratori, come nel caso di migliaia di giovani studenti che intendono lavorare in modo occasionale per mantenersi allo studio famiglie e piccole realtà imprenditoriali che temporaneamente si trovano nell'esigenza di avvalersi di prestazioni di lavoro occasionali senza ricorrere al lavoro nero. Fra le altre misure in tema di lavoro si segnalano quelle relative alla definizione delle caratteristiche che devono avere determinate attività lavorative ai fini della corresponsione dell'indennità riconosciuta, fino alla maturazione dei requisiti pensionistici, a favore di soggetti che si trovino in particolari condizioni (APE sociale), nonché dell'applicazione della riduzione del requisito dell'anzianità contributiva in favore dei cosiddetti lavoratori precoci. Un ulteriore intervento riguarda una modifica alla disciplina sul rilascio del documento unico di regolarità contributiva Relativamente al tema del sostegno alle imprese e ai contribuenti sono state introdotte importanti misure che si articolano in un *mix* di interventi di natura fiscale e di semplificazione

le disposizioni in materia di detassazione dei redditi derivanti da investimenti a lungo termine nel capitale delle imprese effettuati da casse previdenziali e fondi pensione. Tra le misure di sostegno alla crescita si segnalano le nuove disposizioni in materia di agevolazione e di incentivo per gli investimenti in ristrutturazione edilizia. Grazie a queste misure, l'ecobonus si potrà applicare concretamente anche ai grandi condomini sorti negli anni Cinquanta, Sessanta e Settanta, dove le famiglie proprietarie in molti casi sono incapienti. D'ora in poi questo incentivo non servirà soltanto per ristrutturare casa e migliorare l'efficienza energetica degli alloggi delle famiglie che stanno meglio, ma anche degli alloggi posseduti dalle famiglie che finora non hanno potuto beneficiare di tale incentivo. viene molto estesa. La norma ha un enorme potenziale se si tiene conto che nel Paese gran parte dell'ecobonus è stato finora utilizzato per ristrutturare le case singole e, in rarissimi casi, per i grandi condomini. In tema di credito, sono state introdotte importanti misure quali l'estensione dell'ambito di applicazione del Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti e le innovazioni in tema di cartolarizzazione dei crediti. Infine, in tema di investimenti, assumono particolare rilevanza le misure volte all'agevolazione degli investimenti per la realizzazione di importanti eventi sportivi di portata internazionale che devono essere svolti nei prossimi anni nel nostro Paese, nonché le misure di semplificazione degli *iter* procedurali previsti per la costruzione di impianti per le competizioni sportive.

Nel merito, il tema delle Province è stato affrontato tenendo conto che su tali enti è in corso, e sarà oggetto anche nel futuro prossimo, un ripensamento rispetto alla loro collocazione complessiva all'interno dell'ordinamento istituzionale del Paese dopo gli esiti del *referendum* e della loro conferma come enti di rilievo costituzionale. Si tratta di garantire a tali enti la capacità di assolvere pienamente alle funzioni fondamentali importanti che sono loro assegnate, quali quelle in materia di edilizia scolastica, mobilità, viabilità delle strade, tutela dell'ambiente, pianificazione e programmazione, consentendo loro di affrontare al meglio l'attuale fase transitoria ed emergenziale. Con il provvedimento in esame non si risolvono tutti i problemi ancora aperti delle Province, ma si danno prime risposte significative che consentono loro di vivere questa fase di transizione per approdare a un assetto finanziario più stabile e definito, che ha come traguardo il 2019.

Nel frattempo, per gli anni 2017 e 2018 sono state ampliate le risorse a disposizione delle Province fino a 180 milioni di euro per ciascuno dei suddetti per l'esercizio delle funzioni fondamentali, con un significativo incremento rispetto a quanto previsto originariamente dal decreto-legge. Oltre a ciò, sono state approvate altre tre importanti disposizioni. La prima prevede un aumento da 100 a 170 milioni di euro, per il 2017, del contributo in favore delle Province per l'attività di manutenzione straordinaria della rete viaria. La seconda disposizione prevede un'ulteriore autorizzazione di spesa

Come accennato in precedenza, tali misure si aggiungono a quelle originarie che prevedevano, fra l'altro, la ripartizione della riduzione della spesa corrente tra le Province e le Città metropolitane. Analogamente, viene ripartito tra ciascuna Provincia e Città metropolitana il concorso alla finanza pubblica e si prevedono misure per favorire l'approvazione dei bilanci da parte delle Province e delle Città metropolitane per superare la fase di transizione.

Per i restanti Comuni, la percentuale è fissata al 90 per cento. Si segnalano, infine, le disposizioni relative alla determinazione e ripartizione del Fondo di solidarietà comunale e le assai significative misure di semplificazione che discendono dall'entrata in vigore del principio del pareggio di bilancio. vigore del principio del pareggio di bilancio. Per favorire la fusione tra Comuni, è stato previsto che non si applichino nei primi cinque anni della fusione i vincoli stabiliti dalla normativa vigente per le assunzioni a tempo determinato. Per quanto riguarda le Regioni, un'apposita disposizione stabilisce, per l'anno 2017, la ripartizione tra le Regioni a Statuto ordinario degli spazi finanziari per favorire gli investimenti per complessivi 500 milioni di euro, già stanziati dalla legge di bilancio 2017. Un ulteriore intervento riguarda l'attribuzione di quote del Fondo da ripartire per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese.

Nell'ambito del capitolo dedicato agli enti territoriali, sono state introdotte inoltre misure in tema di trasporto pubblico locale e di spesa farmaceutica e sanitaria. al trasporto pubblico locale, si segnala la rideterminazione della consistenza e la definizione dei criteri per la ripartizione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, Inoltre, sono state dettate alcune disposizioni che incidono sulla competitività del settore del trasporto pubblico su gomma, con riferimento ai servizi di linea interregionali con itinerari, prezzi e frequenze prestabilite.

e sui farmaci cui è stato riconosciuto il requisito dell'innovatività condizionata. Ci sono poi altri provvedimenti che troviamo nel testo. Riguardo alla spesa sanitaria si recepisce, con riferimento all'edilizia sanitaria, quanto stabilito dall'intesa Stato-Regioni in merito alla riduzione, pari a 100 milioni di euro, delle risorse programmate per tali interventi nel settore dell'edilizia. Inoltre, sempre con riguardo alla spesa sanitaria, si modifica la norma di deroga che per il 2016 esclude il computo, ai fini della verifica del rispetto dell'obbligo del pareggio di bilancio da parte delle Regioni o delle Province autonome, di alcuni impegni contabili inerenti alla spesa sanitaria. Le misure in favore delle zone colpite dagli eventi sismici rappresentano un altro capitolo di grande rilievo politico e sostanziale del decreto-legge. Fra le misure più significative si ricorda lo stanziamento di un miliardo di euro, per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, per gli interventi previsti nel decreto-legge e l'istituzione di un Fondo per accelerare le attività di ricostruzione,

sismico 1, nonché per specifici piani sperimentali per la difesa sismica degli edifici pubblici e per l'acquisto e la manutenzione dei mezzi occorrenti per il soccorso alla popolazione civile. Gli interventi previsti sono stati ulteriormente ampliati alla Camera, ad iniziare dall'assegnazione di spazi finanziari volti ad agevolare l'effettuazione di investimenti connessi alla ricostruzione da parte degli enti degli enti locali colpiti, misure volte a sostenere le capacità di progettazione dei Comuni nelle aree colpite, misure volte a sostenere ulteriormente le imprese del settore turistico e del commercio, a mettere a disposizione maggiori risorse per la copertura dei cosiddetti danni indiretti derivanti dagli eventi sismici, misure volte inoltre a dare risposta alle istanze presentate dalle imprese agricole relativamente ai danni subiti da eventi calamitosi, non solo per il terremoto, ma anche in relazione ad altri eventi meteorologici quali le gelate.

che si sono susseguiti dal 24 agosto 2016. Ultime, ma non per rilievo, si segnalano le disposizioni in materia di istruzione e di cultura. Per quanto riguarda l'istruzione, è molto importante la norma che aumenta la disponibilità del Fondo destinato all'incremento dell'organico docente e dell'autonomia; un incremento destinato a coprire l'onere per le retribuzioni del personale docente, che si determinerà in conseguenza del consolidamento dell'organico delle scuole di ogni ordine e grado di 15.100 posti provenienti dall'organico di fatto. Si tratta di un investimento di grande importanza, come di grande importanza sono gli interventi sulle istituzioni di alta formazione artistica e sui sistemi bibliotecari locali. Si ricorda inoltre la norma relativa agli incarichi di direttore di istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale, per i quali si afferma un principio: non si costruisce una norma anti-TAR, come erroneamente si è detto, ma si afferma il principio per il quale per il quale i nostri luoghi di cultura ambiscono a poter avere alla loro direzione le migliori professionalità e competenze a livello internazionale. Fra le altre misure, viene incrementato poi di 58 milioni per il 2017 il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili e vi è una serie di altre misure previdenziali e organizzative; ce ne sono alcune che riguardano il potenziamento dell'organico della Corte dei conti, misure sul Fondo per le mense scolastiche biologiche e tante altre iniziative che vanno nel senso di consolidare gli obiettivi e le linee di azione contenuti originariamente nel decreto-legge. si tratta di un provvedimento complesso, importante, che per struttura è paragonabile ai più importanti provvedimenti adottati nel corso di questa legislatura, e a cui è affidato l'obiettivo di allargare il sentiero della crescita

Per quanto riguarda il mio ruolo non mi sento assolutamente offeso dalle sue affermazioni, perché ritengo di interpretarlo sia nella fase politica che nella fase di Presidenza.

è che la nostra Costituzione dovrebbe, finché è in vigore, essere rispettata, indipendentemente dal giudizio che ciascuno ha sulle sue singole parti. Lo impone innanzitutto una ragione etico-morale, essendo la nostra Costituzione la Carta fondamentale che regola la vita della Repubblica. Quando poi si tratta dei rapporti fra lo Stato e le Regioni vi sono anche una ragione di convenienza e una ragione funzionale

La seconda premessa: abbiamo fatto di tutto per non presentare questa questione pregiudiziale. In particolare il collega Di Giacomo, intervenendo nelle sedi proprie di Commissione, ha chiesto a più riprese che

con carattere di necessità e urgenza (quindi con decreto-legge) - del piano operativo straordinario della Regione Molise. Tale piano, concordato attraverso l'intesa Stato-Regione e adottato con decreto del commissario *ad acta*, non è mai stato sottoposto per deliberazione all'organo legislativo della Regione Molise stessa. Come voi sapete, colleghi senatori, l'articolo 117 della nostra Costituzione afferma che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Sempre l'articolo 117, per quanto riguarda le materie concorrenti, tra le quali rientra la sanità, attribuisce alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali riservata alla legislazione dello L'articolo 120 della nostra Costituzione stabilisce poi che il Governo può sostituirsi agli organi delle Regioni in caso di mancato rispetto

Sempre l'articolo 120 dice - e questo mi sembra il punto fondamentale - che la legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di leale collaborazione. colleghi senatori, la giurisprudenza costituzionale ha stabilito che l'autonomia legislativa delle Regioni in materia di tutela della salute possa subire limitazioni, ma ha aggiunto che queste devono comunque essere circoscritte a iniziative legislative o attività di delegificazione da parte del Consiglio regionale al fine del rispetto dell'attuazione del piano di rientro. Inoltre, sempre la giurisprudenza costituzionale ha stabilito che il legislatore nazionale può intervenire in caso di dissesto finanziario solo attraverso la fissazione di limiti complessivi alla spesa, lasciando al livello di governo locale o regionale «ampia libertà di allocazione delle risorse fra i diversi ambiti e obiettivi di spesa» (secondo la sentenza n. 415 del 2005

È possibile porre limiti; non è possibile estromettere completamente l'organo legislativo della Regione da questa procedura.

del principio di leale collaborazione fissato dalla Costituzione passiamo all'istituzione di un principio di leale sostituzione da parte dello Stato. Se poi leggiamo sugli organi di stampa le reazioni provocate da questo provvedimento nella Regione interessata, dobbiamo concludere che il principio non è di leale sostituzione, ma di sleale sostituzione, perché evidentemente il Consiglio e e l'organo legislativo vengono completamente estromessi. A me pare, signor Presidente e colleghi, che si stia stabilendo un precedente o quantomeno si stia consolidando una prassi che rischia di creare un contenzioso foriero foriero di nuovi problemi e ritardi. Al di là delle intenzioni, che possono essere anche eccellenti, poiché sappiamo che di buone intenzioni è lastricata la via dell'inferno dovremmo tener presente tutto ciò, soprattutto quando si tratta della Costituzione

Signor Presidente, per l'ennesima volta dobbiamo sollevare le medesime eccezioni e considerazioni già svolte in altre sedi nel momento in cui sono stati emanati decreti-legge in mancanza totale dei presupposti previsti dalla Costituzione.

dalle sentenze della Corte costituzionale. Ricordo, a tacer le altre, la ormai più volte citata nelle pregiudiziali di costituzionalità che abbiamo proposto in molte altre sedi, la sentenza n. 171 del 2007.

gli unici presupposti veramente fondanti per l'emanazione del decreto-legge in esame potrebbero riguardare le misure per la tutela delle popolazioni colpite dagli eventi sismici. Questo sì.

Per quanto riguarda comunque la tutela delle zone colpite da eventi sismici, vi è stata una pluralità di normative, di richiami legislativi, di proroghe, di rinvii,

il contenuto del decreto-legge deve essere «specifico, omogeneo e corrispondente al titolo». Immancabilmente ci ritroviamo, invece, con un provvedimento che comprende normative tra di loro molto diverse. Ricordiamo, oltre alla finanza pubblica, interventi in materia di giustizia tributaria, contenimento della spesa pubblica, disposizioni in materia di enti territoriali, trasporti e infrastrutture; e poi arriviamo a misure per il lavoro, la produttività delle imprese, interventi per eventi sportivi e in materia di servizi. Quindi, vengono trattate più materie nello stesso provvedimento,

Facciamo un esempio: l'articolo 1 prevede l'emanazione di un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze per l'attuazione delle nuove misure per il contrasto fiscale in materia di *split payment*. Inoltre, all'articolo 4, un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate per l'attuazione delle nuove misure di regime fiscale per le locazioni brevi. Dunque, anche in questo caso si disattende la portata e quello che dovrebbe essere il contenuto

payment*, applicato a tutte le amministrazioni, enti e soggetti inclusi nel conto consolidato della pubblica amministrazione, nonché ai liberi professionisti. Anche in questo caso, cogliamo l'occasione

enti, associazioni e professionisti che avranno problemi di liquidità. È una questione che è già stata sollevata più volte

pertanto, avrebbe ben potuto, oltre che dovuto, varare la manovra con quattro mesi di anticipo senza ricorrere, *in extremis*, alla decretazione d'urgenza e consentendo al Parlamento di esercitare pienamente le sue prerogative istituzionali;

di tali requisiti doveva essere, infatti, rilevabile non soltanto nel preambolo e doveva essere, come al solito, sostanziale. Quindi, da questo punto di vista ci troviamo di fronte a un decreto che,

67, da questo punto di vista non hanno alcuna connessione logica tra di loro e neanche con la manovrina. Quindi, con decreto *omnibus*, il Governo ancora una volta ha disatteso il monito a una maggiore attenzione al profilo della omogeneità di contenuto dei decreti-legge, decreti-legge, più volte lanciatogli dalla Corte costituzionale; per la quale Corte la non omogeneità del contenuto di un decreto-legge rappresenterebbe un indice, o meglio un indizio, assolutamente certo della insussistenza del requisito della straordinaria necessità e urgenza.

Grazie.

confronto con i cittadini e ha dunque pensato non di modificare, ma di abrogare la norma, in modo tale che la Corte di cassazione, tra l'altro, non si dovesse neanche pronunciare.

petrolifere all'interno delle 12 miglia. Non è tollerabile che un Governo metta in campo operazioni di aggiramento delle norme che sono a garanzia di tutti

Si è prodotto uno strappo fortissimo nei confronti della democrazia, essendo tra l'altro, anche

Vi sono poi altre due questioni molto rilevanti, dal punto di vista costituzionale. Mi riferisco all'articolo 62, in cui peraltro si interviene per facilitare

della Regione Molise: si fa un'operazione molto grave che apre il varco alla privatizzazione della sanità molisana, declassa l'ospedale pubblico, non garantisce i LEA e sancisce il principio che un piano sanitario può essere approvato dal Parlamento e non dal consiglio, espropriando completamente in quel caso i consigli comunali e, in questo caso, i consigli regionali di competenze proprie. Per tutti questi motivi, signor Presidente, chiediamo a quest'Assemblea, anche per respingere

cercherò di non intrattenere eccessivamente quest'Assemblea con i temi di legittimità costituzionale che sono stati già indicati e ampiamente argomentati dai colleghi che mi hanno preceduto, ma purtroppo questo è un intervento che dobbiamo ritualmente ripetere sia in Commissione che in e lo dico con profondo sconforto. Noi abbiamo un vaglio di costituzionalità che parte dalla Commissione affari costituzionali e si basa principalmente, per quanto riguarda i decreti-legge, sulla compatibilità con l'articolo 77 della Costituzione. Come voi tutti mi insegnate,

primaria) cause, motivi, ragioni conclamate ed evidenti di necessità e urgenza. Richiamo inoltre un articolo della legge n. 400 del 1988, che ormai abbiamo talmente tanto evocato in quest'Aula che, se ognuno di noi fosse in grado di ricevere un euro per ogni evocazione, sarebbe ricco.

Grazie. che hanno come ambito di applicazione l'universo mondo. Si va dalla materia fiscale alla materia di lavoro, alla materia immobiliare, alle procedure di insolvenza, a questioni notoriamente necessarie e urgenti come interventi sulla tratta Salerno-Reggio Calabria - quindi, una necessità e urgenza che va avanti da circa una cinquantina di anni materie che attengono ad ANAS, alle Ferrovie dello Stato, alla regolamentazione di settori della pubblica amministrazione. E faccio tutti questi riferimenti, perché questa norma evidentemente non è necessaria né urgente,

le calamità naturali, ma anche in quel caso ho seri dubbi. Né tantomeno si può parlare di omogeneità. Il vero unico e grande filo conduttore del provvedimento è rimediare alla legislazione sciatta, disorganica e affastellata che ha caratterizzato i mille giorni di Governo Renzi e che purtroppo questo Governo sta terribilmente continuando. Un esempio ne è la materia fiscale. Abbiamo avvertito il Governo e la maggioranza che lo sostiene che il decreto fiscale approvato con i voti di maggioranza - lo sottolineo - al chiudersi dello scorso anno anno identificava problemi e patologie per gli operatori del settore e, soprattutto, per i destinatari della norma molto rilevanti. Questa manovra, tra l'universo mondo di materie che sta regolamentando, tenta di risolvere - ahimè invano, perché stiamo accumulando errori su errori - problemi problemi determinati da una legislazione fiscale precedente sempre attuata per decreto - costituisce una patologia nella patologia della patologia - che ha creato grosse difficoltà attuative.

Un altro esempio la materia dei *voucher*. Il tanto conclamato e sbandierato *jobs act* ha creato problemi immensi al mercato del lavoro e continuerà, purtroppo, a crearne, posto che una buona parte della droga Il settore dei *voucher* - lo hanno ricordato i colleghi che mi hanno preceduto trattato in maniera manichea e tranciante con un colpo di ascia, che rappresenta in se stesso un margine di incostituzionalità, obliterando una richiesta di *referendum* supportata dalla raccolta di firme di cittadini che quel *referendum* chiedevano. Ancora una volta, in maniera arrogante e incospicua, il Governo, senza consultare alcuno e identificare dei centri di interesse nella rappresentanza di categoria e identificando solo in se stesso il centro di imputazione della ragione o del torto, ha cancellato uno strumento indispensabile per le famiglie, per le imprese, per gli artigiani e i commercianti, non elaborando alternative. All'interno del provvedimento in esame si tenta di elaborare alternative che, dal momento che una parte di noi ritiene identiche

Ciò che dovrà sostituire i *voucher* non servirà e sarà più oneroso per le famiglie e insufficiente per le imprese, gli artigiani, i ristoratori, per il settore del turismo e il comparto dell'agricoltura. La misura non basterà a ridare quello che è stato ingiustamente tolto sotto il profilo sia del merito e dei contenuti,

Un esempio riguarda il settore del trasporto pubblico locale. L'articolo 27 interviene sul fondo che regolamenta l'alimentazione del trasporto pubblico locale, aumentandone l'entità e

intese non ci sono. Oltre agli elementi di incostituzionalità relativi alle competenze concorrenti tra Stato e Regioni identificati dai colleghi che mi hanno preceduto, nuovi margini di incostituzionalità ricadono quindi sul provvedimento

ognuno di noi sa o dovrebbe sapere che, quando si tratta di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, il diritto di stabilimento non vale, salvo deroga. Perché questo Governo, ancora una volta in maniera sciatta, si è sottoposto all'umiliazione di vedersi annullare delle nomine dal tribunale amministrativo regionale? E, soprattutto, come può pensare che questa patologia venga sanata all'interno di un decreto-legge disomogeneo senza violare chiari parametri di costituzionalità?

non ha consolidato i conti pubblici e non ha attuato quella semplificazione che da anni - cioè dall'inizio del Governo che ha preceduto l'attuale, rispetto al quale quest'ultimo si muove in continuità - viene promessa

Non compiacciamoci dell'aumento captato dal Fondo monetario internazionale: un aumento minimo che, purtroppo, sarà controbilanciato dal rischio di forti *shock* negli anni a venire. Questa manovrina non serve. Tutto quello che è stato fatto - ripeto - in spregio alla Costituzione non produrrà purtroppo alcun effetto. È per questo motivo che noi chiediamo che il provvedimento fermi in questo stadio il suo percorso in quest'Aula parlamentare.

Presidente, prendo la parola per il Gruppo Articolo 1-Movimento Democratico e Progressista e anticipo già che voteremo contro le pregiudiziali. Ma abbiamo bisogno di intervenire nella discussione, perché comunque vogliamo segnare una differenza. ci sono degli elementi critici che abbiamo a più riprese portato avanti nei luoghi a ciò deputati, nelle Commissioni, e anche nei luoghi politici: questo è il luogo giusto per ribadirli,

non potremmo dolerci di nulla. Tra l'altro, non è stata introdotta nemmeno con il decreto-legge n. 50 del 24 aprile 2017, che oggi l'Atto Senato 2853 converte in legge.

il Governo sembrerebbe infatti trovarsi nella posizione di chi non ha fatto nulla di particolarmente grave, se non fosse che gli emendamenti molto spesso vengono presentati nelle Aule anche su sollecitazione del Governo e comunque vengono approvati con il parere il tema c'è, in tutta la sua gravità, e si pone. Perché si pone questo tema? Ci siamo trovati davanti a una normativa sui *voucher* che ha sollecitato molti contrasti anche all'esterno del palazzo e su cui è stato presentato un *referendum* che

il 21 aprile, un'ordinanza con cui ha sospeso la procedura del *referendum*. Sono state diramate le varie circolari sul territorio e di fatto il *referendum* non si è tenuto e non si può più tenere. Immediatamente dopo, però, la Camera ha introdotto una normativa che, se non è quella dei *voucher*, è molto simile. È troppo facile dire che non è quella, perché non c'è il termine o perché è leggermente diversa;

sentenza n. 68 del 1978, che avrebbe consentito alla Cassazione di verificare se il *referendum* dovesse essere trasferito sulla nuova normativa, oppure se non si dovesse dare luogo al *referendum*. Invece, si chiude l'argomento *referendum* e se ne apre un altro: una nuova normativa su cui eventualmente si dovranno raccogliere nuove firme. Tutto questo non ci sembra democratico e a ben vedere non è nemmeno corretto sul piano procedurale. Il punto è di chi sia la competenza a sollevare tale questione. Per questo non abbiamo presentato una questione

oggi contestando questa procedura, sicuramente non lineare. Sarà allora probabilmente il comitato promotore a dover sollevare la questione, con l'unico strumento che intravedo, quello del conflitto di attribuzione. Sarà probabilmente la Corte costituzionale che potrà, in via incidentale, sollevare una

perché quando si è intervenuti su norme, su cui era stato ammesso il *referendum*, per modificarle, la Cassazione ha potuto dire sì o no, è sufficiente o non è sufficiente per eliminare il *referendum*, mentre in questo caso si è aggirata una procedura. Tutto questo dunque comporta l'incostituzionalità e pone un problema politico enorme su un argomento che, tra l'altro - come qualcuno ha detto poco fa - dovrebbe essere oggetto di concertazione e dibattito, soprattutto quando una sigla sindacale ha raccolto

con metodi democratici, portano avanti con una firma per un *referendum*: un metodo democratico con cui si porta avanti un'opinione. Tutto questo però non ci porta oggi a votare a favore della questione pregiudiziale, perché siamo consapevoli dei compiti che ha il legislatore:

a superarle, anche quelle che, per la verità, non sono di poco conto, a prescindere dalla costituzionalità: parlo di merito. Ma sui *voucher* tutto questo non è possibile. Sui *voucher* c'è un *vulnus* molto grave che ha

Signor Presidente, mi rallegro del fatto che sia proprio lei a presiedere in questo momento. non avevo previsto un mio intervento su questo tema perché avevamo demandato, come sempre facciamo, alla Commissione competente il

Abbiamo già iniziato a parlare di questioni di fiducia e qualcuno - anche lei - ha detto che è quasi un atto dovuto.

vuole abbandonare l'Aula di farlo in silenzio, per consentire al senatore Lucidi di svolgere il suo intervento. LUCIDI *(M5S)*. Vorrei semplicemente segnalarle quanto sta avvenendo in queste ore. Noi abbiamo abbiamo accolto questo provvedimento enorme, come ha detto il relatore Santini, definendolo addirittura «un sentiero stretto»; in realtà, noi riteniamo che, più che un sentiero stretto, questo sia un vero eproprio *cul-de-sac*, perché è proprio lì che siete andati a finire con questa maggioranza. Non so se lei lo sappia, caro Presidente, ma ieri è stato votato un parere negativo in Commissione affari esteri: la maggioranza non la maggioranza non è riuscita ad esprimere un parere positivo su quanto era stato portato in Commissione dal relatore Sangalli.

che, addirittura, questa mattina la Commissione ambiente non sono riuscite a deliberare quel parere che la maggioranza, invece, aveva portato in Assemblea. Detto questo, riteniamo che sia invece un passaggio fondamentale.

ancora una volta, le nostre prerogative costituzionali e, in questo caso, l'importanza del lavoro in Commissione sono stati assolutamente scavalcati. Alcuni articoli del nostro Regolamento

Grazie

Come gli italiani, anche le Commissioni sono ostaggio delle pulsioni elettorali di un ex Presidente del Consiglio totalmente delegittimato*. Signor Presidente, innanzi tutto credo dobbiamo porci una domanda rispetto a questo decreto-legge, che non sta semplicemente nel valutarne i contenuti, ma nel chiedersi perché è necessaria una manovra correttiva. risposta sia facile: la manovra correttiva si è resa necessaria perché l'ultima legge finanziaria del Governo Renzi era un'evidente manovra propagandistica, che conteneva interventi senza alcuna copertura,

pressoché incontrastato per i prossimi anni. Ebbene, i risultati li abbiamo visti tutti: nonostante la manovra elettorale, Renzi è stato sonoramente sconfitto dagli elettori e mandato a casa. Ovviamente, il compito di mettere insieme i cocci e di mettere ordine nei conti pubblici è toccato al Governo Gentiloni che sta adottando in questa manovra vecchi metodi, che non sono assolutamente quelli necessari alla crescita economica del Paese. Paese. S'intende sostanzialmente mettere ordine nei conti pubblici dissestati dal Governo Renzi con un intervento che si può quantificare in 3,1 miliardi di euro, composto quasi esclusivamente dall'aumento della pressione fiscale, dall'aumento della pressione fiscale, che arriva a rappresentare quasi 3 miliardi di questa manovra. È quindi difficile poter parlare di misure per il rilancio economico e lo sviluppo, come questo

Gli aumenti di prelievo si riferiscono ad esempio allo strumento dello *split payment*, attraverso il quale si è già fatto abbastanza danno alle imprese

le agevolazioni per le imprese; di fatto, aumentando la base imponibile, si aumentano le tasse per le imprese. Si tratta anche in tal caso di un provvedimento di prelievo fiscale ad un sistema produttivo che invece avrebbe bisogno di agevolazioni e non certo di nuovi carichi fiscali.

dell'impatto delle clausole di salvaguardia, che in realtà è assolutamente minimale: acquisire dall'aumento dell'IVA e dall'aumento delle accise, c'è una riduzione esclusivamente parziale. Dopo cinque anni - al termine di una legislatura partita con queste clausole presenti, perché l'aumento dell'IVA e delle accise sulla benzina saranno

della propria attività legislativa, non riesce ad annullarle e sterilizzarle, e si limita a rinviarne ulteriormente l'applicazione.

con episodi raccapriccianti, come il sorteggio delle abitazioni provvisorie. Ebbene, c'è sempre una rincorsa a risolvere le emergenze con mesi o anni di ritardo. L'avevamo denunciato fin dall'inizio attraverso gli interventi dei colleghi colleghi Arrigoni e Candiani e ora i nodi arrivano al pettine. Arrivano i nodi, con provvedimenti tardivi, probabilmente non risolutivi, con grave colpevolezza nei confronti di persone che si trovano in una situazione di grave emergenza. Questi sono solo alcuni temi, ma ve ne sono molto altri negativi in un provvedimento che alla fine rappresenta un tentativo maldestro di correggere i gravi errori e le gravi responsabilità dell'ultimo Governo del presidente

In questo provvedimento vi è uno stanziamento per la statizzazione di 18 istituti musicali *ex* pareggiati e delle 5 accademie storiche. di una misura lungamente attesa da parte di questi istituti che si sono trovati, loro malgrado, in condizioni finanziarie tragiche

che hanno permesso loro di galleggiare in un regime di transitorietà, di precarietà, di mera sussistenza che poco si addice addice a degli autentici presidi culturali in territori anche difficili: penso ad esempio ad alcuni istituti della Sicilia, Regione da cui provengo.

possono essere davvero un punto di partenza per la rinascita del territorio. Ebbene, tutto questo è stato mortificato, è stato in qualche modo penalizzato da una politica assolutamente miope

che hanno permesso a questo e ad altri istituti di galleggiare ma che sostanzialmente ratificano, ancora una volta, una visione miope della politica culturale di questo Governo. Con questa manovra, noi ci troviamo di fronte a quella che dovrebbe essere - sottolineo dovrebbe essere perché è ancora da dimostrare che lo sia - la tanto auspicata e finale statizzazione. Dico dovrebbe esserlo innanzitutto perché le risorse sono del tutto insufficienti per una completa statizzazione di tutti gli istituti, perché il processo di statizzazione viene demandato ad un successivo decreto ministeriale e noi, naturalmente, sappiamo che in questo campo - ahimè - la storia dei decreti attuativi delle leggi

Una politica culturale fatta in questo modo, secondo me, non è degna di un Paese civile, di un Paese che vorrebbe ripartire e che dovrebbe ripartire proprio da questi settori.

accantonato grazie al consistente contributo statale di cui questa fondazione di diritto privato ha usufruito. Soldi stanziati e inutilizzati, che l'IIT non ha saputo sfruttare proprio a causa dell'ingente finanziamento di cui ha goduto, a differenza delle università e degli enti di ricerca, che invece hanno sofferto

saranno usati dall'Istituto di tecnologia che - pensate - assurgerà al rango di vera e propria agenzia pubblica di finanziamento: una autentica stortura, contro la quale bisognerebbe urlare e ergersi, perché si sta dando a una fondazione di diritto privato addirittura la potestà di agenzia di finanziamento di soldi pubblici ricevuti.

pare, signor Presidente

la cosiddetta manovrina recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria», provvedimento molto importante, che comporta interventi correttivi sui conti pubblici per il 2017 pari a 3,1 miliardi, con un effetto migliorativo di circa 0,2 punti percentuali di PIL, è frutto di una correzione già prefigurata nel DEF 2017, sulla base di accordi intercorsi tra Governo e Commissione europea. Ritengo assolutamente soddisfacente questa serie di interventi, molteplici interventi, molteplici e definiti in maniera molto precisa dalla relazione del senatore Giorgio Santini: dall'estensione dell'ambito applicativo dello *split payment*, speciale meccanismo di versamento dell'IVA introdotto dalla legge di stabilità 2015, applicato nei rapporti tra imprese private e pubblica amministrazione, secondo il classico meccanismo dei pagamenti divisi; alla cosiddetta *web tax*, ovvero alle società multinazionali non residenti con ricavi superiori ad un miliardo di euro, alle modifiche alla disciplina della riapertura dei termini per quanto riguarda la collaborazione volontaria in materia fiscale, la cosiddetta *voluntary disclosure*. Per procedere, poi, con varie misure come quelle di contrasto alle compensazioni fiscali indebite, all'incremento delle tassazioni sui tabacchi e sui giochi, all'inibizione dei siti *web* recanti offerte di alcuni prodotti da tabacchi o pubblicità di giochi e scommesse. Tra le misure che interessano il settore della finanza locale, abbiamo le disposizioni in materia di enti territoriali che recano la concessione di contributi nei confronti di Province, Città Metropolitane e Regioni a Statuto ordinario. Tra l'altro, sono fondamentali anche le disposizioni che si introducono volte all'agevolazione dell'approvazione dei bilanci da parte di Province e delle stesse Città metropolitane e atte a modificare alcune scadenze per gli enti dichiarati in dissesto. Tra le varie disposizioni e misure della cosiddetta manovrina, vorrei evidenziare la positività di quelle urgenti afferenti alle zone colpite dai recenti eventi sismici, in favore delle quali vengono stanziati tre miliardi per il triennio 2017-2019 e viene istituito un Fondo per accelerare le attività di ricostruzione. Ritengo assolutamente positiva, inoltre, la previsione di ulteriori interventi agevolativi fiscali: in particolare, la proroga dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari o la

decisamente apprezzabile la prevista assegnazione di finanziamenti finalizzati ad agevolare investimenti nei territori colpiti dagli eventi sismici rivolti alle imprese del settore turistico-commerciale, ma anche favorenti la ripresa

Tutto ciò mi induce ad auspicare fortemente che le zone franche urbane, o le zone economiche speciali (ZES), vengano istituite, come già avviene in taluni Stati membri dell'Unione europea, anche per altre aree particolarmente depresse del Paese, oltre a quelle colpite dai gravissimi eventi calamitosi, specie quelle confinarie e che risentono di svantaggi derivanti da differenti livelli di imposizione fiscale tra Paesi contigui.

all'attrazione di investimenti produttivi anche esteri, al rilancio del tessuto produttivo, dell'occupazione, della competitività e dello sviluppo dei territori di riferimento. Obiettivo delle ZES delle ZES è ridurre il regime impositivo, al fine di agevolare una rapida crescita economica delle zone interessate.

oggi presentano una situazione di particolare difficoltà economica e produttiva, in particolare nelle aree di confine dello Stato

Auspico che il Governo si impegni ad aprire un tavolo di confronto con l'Unione europea al fine di valutare le procedure e le modalità per la realizzazione, anche nel nostro Paese, in determinate aree territoriali che presentano una situazione di difficoltà produttiva o che subiscono, anche in ragione della prossimità territoriale con altri Stati, svantaggi competitivi derivanti

(non eravamo abituati a votare i provvedimenti di questo Governo e di questa maggioranza che hanno cancellato ogni forma di diritto nel mondo del lavoro), ma lo avremmo fatto perché era frutto di una lotta, frutto di democrazia. Ricordo che la CGIL aveva raccolto 3,5 milioni di firme per quel *referendum* e quindi per tutti questi motivi avevamo votato quel provvedimento.

e quando lei ha detto che la trasparenza dei nuovi *voucher* - così ha detto - farà emergere il lavoro nero, devo dirle con profondo rispetto che lei non ha letto il provvedimento in esame, altrimenti dice cose non vere.

«È vietato il ricorso al contratto di prestazione occasionale: *a)* da parte degli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato». Non si capisce bene da dove arrivi questa norma, ma le dico cosa succederà,

Guardate bene cosa dite al punto 18: «Nel caso in cui la prestazione lavorativa non abbia luogo, l'utilizzatore di cui al comma 6, lettera *b)*, è tenuto a comunicare, attraverso la piattaforma informatica INPS ovvero avvalendosi dei servizi *contact center* messi a disposizione disposizione dall'INPS, la revoca della dichiarazione trasmessa dall'INPS entro i tre giorni successivi». Così emerge il lavoro nero? Non so veramente di cosa state parlando.

abbiamo sempre detto che di voi non ci fidiamo. I fatti sono sotto gli occhi di tutti. Se vi serve un provvedimento di questa natura per dire che la disoccupazione è scesa dello 0,01 siete proprio fuori strada perché il provvedimento può servire solo a una cosa del genere perché non parliamo di lavoro. Ricordo a tutti, poiché sembra che prima dei *voucher* questo tipo di lavoro non esistesse,

Signor Presidente, Vice Ministro, onorevoli senatori, il testo del decreto-legge, che non ci è consentito modificare, mortifica a mio avviso il ruolo del Senato, quasi che la riforma costituzionale fosse stata approvata e quest'Aula abolita. Eppure siamo davanti a una manovra di aggiustamento dei conti pubblici che di norma richiede l'esame di entrambi i rami del Parlamento. Tra l'altro, si tratta di un manovra con più di 130 articoli che trattano una varietà di temi e argomenti. Insomma, un provvedimento *omnibus* che alla Camera, ogni giorno che passava, si ingrandiva di nuove materie e commi. Quando si parla di manovra, manovrina, punti di *deficit*, aggiustamento di conti spesso

credo che quando si dice che si riduce di 0,2 punti il *deficit*, portandolo dal 2,3 al 2,1, si saranno chiesti cosa significa. Ebbene, cari cittadini, significa che si aumentano le tasse, perché questa manovra è fatta per 2.921 milioni di nuove entrate e solo per 181 milioni di riduzione della spesa. Non solo, aggiungo che le maggiori entrate derivano da meccanismi di calcolo di gettito dell'IVA, *split payment*, compensazioni e detrazioni che penalizzano imprese e liberi professionisti. Insomma, il Governo invece di favorire chi in questo Paese produce e lavora, cerca di contrastarlo in ogni modo. Per il terremoto del Centro Italia non vi sono somme aggiuntive per l'anno in corso e quelle previste per il prossimo anno, pari a 885 milioni di euro, hanno coperture che andranno confermate a fine anno dalla legge di bilancio e che, comunque, sono di gran lunga inferiori ai miliardi di euro che ogni anno

ha messo in questo provvedimento di tutto e di più, senza un criterio logico e una prospettiva, cercando di assecondare, o far finta di assecondare, le richieste dell'Europa, che ci ha ammonito per il *deficit* eccessivo. una storia già vista, con un finale già visto: un provvedimento che mette una toppa e, soprattutto, mette le mani nelle tasche degli italiani, delle famiglie e - perdonatemi - delle piccole imprese. Ho parlato di maggioranza di Governo, ma in realtà dovrei parlare di maggioranze di Governo. Pensiamo, ad esempio, al tema dei *voucher*, dove si è scatenata una battaglia senza esclusione di colpi nella sinistra, che ha perso di vista la realtà del problema e si è focalizzata invece su argomentazioni ideologiche e dogmatiche. Ebbene, se la sinistra esterna e interna al Partito Democratico vuol far cadere il Governo è liberissima di farlo, ma non si prendano a pretesto i *voucher*. Non si può utilizzare un tema così serio e importante come causa di una caduta di Governo. i *voucher* sono indispensabili e costituiscono un'opportunità sia per i lavoratori, che per le imprese. Chi finge di non capirlo è in malafede, o non conosce per niente il mondo dell'impresa, né quello del lavoro. Come accennavo, in alcuni settori, come ad esempio quelli del turismo e dell'agricoltura, l'utilizzo dei *voucher* per la regolarizzazione del lavoro precario e l'emersione di quello sommerso è utile, anzi necessario, perché si tratta di settori che si caratterizzano per prestazioni di lavoro occasionali. Occorre quindi sgombrare il dibattito da pregiudizi ideologici e guardare seriamente alle necessità reali. L'abolizione dei *voucher* è stata un errore. Bisogna rimediare subito, perché altrimenti si arreca un danno significativo a migliaia di lavoratori e a tutti gli imprenditori, soprattutto quelli minori, che facevano un uso virtuoso dei *voucher,* portando a galla il lavoro in nero e offrendo possibilità di occupazione, seppur temporanea, a chi in mancanza dei buoni non poteva accedere al mercato del lavoro. Altra cosa, invece, è l'uso perverso che - ahimè - c'è stato dello strumento da parte di qualcuno, ma, come si suol dire, bisognava evitare di buttare il bambino con tutta l'acqua sporca. è stato pubblicato dall'ISTAT il Bilancio demografico nazionale. L'anno scorso quasi 115.000 nostri concittadini hanno lasciato l'Italia per andare a cercare una vita migliore in altri Paesi. 12.000 persone in più rispetto al 2015. Non solo, continua lo spopolamento del Sud, con un flusso ininterrotto di nostri giovani, e meno giovani,

Per sostituire i vecchi *voucher* avete introdotto, per le famiglie, il libretto famiglia e, per le aziende, il nuovo contratto di prestazione occasionale. Vedremo alla prova dei fatti se questi strumenti, che al momento appaiono confusi anche per noi addetti ai lavori, risulteranno utili o no. Tuttavia, un Governo diligente non può andare alla cieca varando provvedimenti le cui conseguenze sono imprevedibili. In conclusione, onorevoli senatori, Vice Ministro, membri del Governo, secondo noi sono mancati - ahimè - il coraggio di risposte strutturali ai problemi degli italiani e quella concretezza che chiedevamo e auspicavamo per le famiglie e le imprese italiane.

rinunciato a fare questo intervento, perché a quasi un anno di distanza un nuovo incidente, ancora in Puglia, sulle linee delle Ferrovie del Sud-Est, pone nuovamente al centro il tema della sicurezza, che purtroppo nemmeno il clamore della tragedia e le vittime dello scorso luglio sono riuscite a garantire e irreggimentare. Tra treni che ripartono senza velocità sporchi, come nel caso da me denunciato ieri di un Frecciargento partito da Lecce in condizioni vergognose, fotografate dai passeggeri (e non sono accettabili né sufficienti le giustificazioni che lo indicano entrato in sostituzione all'ultimo minuto di una vettura guasta), e il rischio di sicurezza che tracima vergognosamente le percentuali minime prevista dalla statistica, beh, credo che questo complesso, affastellato e articolato problema delle ferrovie del Salento e della Puglia

che cammina su una rete a binario unico, con il rischio intollerabile di morire perché c'è la possibilità che due di questi treni si scontrino fronte a fronte, non appartiene in alcun modo alla logistica contemporanea. Chiedo pertanto per suo tramite, signor Presidente, che il Ministro competente venga a riferire sulle iniziative straordinarie che il Governo intende assumere. che il Governo è da mesi il proprietario delle Ferrovie del Sud-Est. Qualche mese fa, subito dopo la tragedia del luglio scorso, mi feci anche ispiratore di un disegno di legge che poneva il tema della sicurezza e che chiedeva di assoggettare allo stesso organismo di controllo e agli stessi livelli le ferrovie date in concessione e le ferrovie appartenenti direttamente alla rete nazionale;

mai più morti annunciate, speriamo. Bene hanno fatto i magistrati di Messina a condannare la procura di Caltagirone per non aver protetto, nel 2007, Marianna Manduca dalla violenza omicida del marito Saverio Nolfo, nonostante le 12 denunce cadute nel vuoto. È la stessa condanna che aveva rivolto all'Italia la Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo, nel marzo di quest'anno, per il caso Talpis.

È morto poi il figlio, per mano del marito, mentre la signora Talpis ha subìto una coltellata. Per questo ancora una volta, per la mancata protezione

per il lavoro che insieme stiamo portando avanti - sta emergendo come uno dei temi cruciali sia proprio quello della protezione efficace delle vittime ad alto rischio.

Unito ad ogni femminicidio segue una *domestic homicide review*, ovvero un'analisi attenta e dettagliata dei fatti, per capire quale sia stato l'anello debole della rete di protezione che non ha funzionato. Quindi una buona pratica anche questa, che può essere adottata dal nostro Paese e finalmente i magistrati di Messina sono stati antesignani in questa direzione. Ma gli orfani della signora Manduca hanno bisogno di protezione. Per questa ragione voglio davvero sollecitare la Commissione giustizia a portare presto in Aula il disegno di legge per gli orfani dei femminicidi. Quindi, anche da questo provvedimento, che è nelle mani del Senato della Repubblica, può arrivare per tutte le vittime una nuova speranza. in particolare sollecitiamo in tutto il Paese per un radicale cambiamento e l'eliminazione di questa grave forma di violazione di diritti umani richiamare ciascuno ad assumersi la propria responsabilità: magistrati, operatori delle Forze dell'ordine e dei servizi sociali. Ciascuno deve ascoltare con grande attenzione, non solo le denunce, ma anche quel grande sommerso di sofferenza che patiscono moltissime donne vittime della violenza domestica. apre una nuova finestra"). Dichiaro chiusa la votazione a scrutinio segreto per l'elezione di un componente del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti. Ai sensi dell'articolo 25, comma 2, del Regolamento, invito tre senatori Segretari a procedere allo spoglio delle schede e al computo dei voti. *Hanno preso